onorevoli colleghi, il concetto di autonomia universitaria, così come perfezionato dal centrosinistra nel lontano 1999, è diventato ormai sinonimo di irresponsabilità. Irresponsabilità finanziaria e gestionale, a sua volta causa ed effetto di un'irresponsabilità accademica e persino didattica, com'è testimoniato dal costoso proliferare di corsi assurdi e inutili. Non c'è bisogno infatti di ricordare che in Italia - il Paese europeo con il più basso tasso di laureati nella fascia d'età tra i 25 e 34 anni esistono organigrammi di facoltà che talvolta coincidono con alberi genealogici, atenei in cui la qualità della produzione scientifica di alcuni docenti è difficile da valutare in quanto assente, mentre gli studenti sono alle prese con insegnamenti di dubbia utilità formativa, proliferati per mere esigenze politiche se non addirittura familistiche. Di fronte ad una simile idea di autonomia - una autonomia senza responsabilità, l'autonomia dei bilanci in rosso e dei concorsi aggiustati - la riforma del ministro Gelmini risponde in maniera pragmatica ed incisiva ad almeno tre interrogativi che la politica ha il dovere di rivolgere al composito mondo dell'università italiana, e cioè: possiamo permetterci di continuare a finanziare un sistema senza valutare la qualità di ciò che produce? produce? È pensabile che in tempi di crisi economica il nostro Paese moltiplichi scriteriatamente le sedi universitarie per soddisfare semplici interessi campanilistici? Infine, è giusto che i molti professori che fanno ricerca e didattica di alto livello vengano pagati quanto altri professori (non molti, ma comunque troppi) che non fanno nulla? Certamente no. Ed allora ben vengano le novità introdotte da questo provvedimento: dal sistema di valutazione dei risultati per poter allocare le risorse anche in base al merito e alla qualità della didattica al sorteggio delle commissioni di concorso; dall'incentivazione alla federazione di più università per razionalizzare la distribuzione delle sedi, al fondo per il merito, destinato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti. E ben venga, infine, il potenziamento funzionale dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università che, con questo disegno di legge, mira a rivestire un ruolo cruciale nell'implementazione della riforma, sia presso il corpo docente che nei confronti degli studenti. di riforma del sistema universitario, e prima ancora dell'istruzione pubblica, formulata dal ministro Gelmini e dalla stessa portata avanti con convinzione e coraggio in questi anni, certi suoi detrattori - prima i professori, poi gli studenti, ora i ricercatori - hanno sempre invariabilmente opposto la questione della riduzione delle risorse pubbliche quale elemento di scontro frontale, a prescindere da qualsiasi discorso sui contenuti. E l'opposizione, rifiutando il confronto in Commissione, ha purtroppo, a mio avviso, sposato in una linea che mira a rimandare e a strumentalizzare, piuttosto che ad affrontare la questione del rinnovamento dell'università. I tagli - che per il 2011 verranno peraltro in parte ripianati dal Governo -rappresentano infatti troppo spesso un alibi e le preoccupazioni sul futuro dei giovani e del Paese finiscono con l'essere fantasmi agitati per pura convenienza politica. L'università italiana ha bisogno di una rivoluzione etica, capace di generare gestioni economiche sostenibili e proposte formative che vadano oltre l'autoreferenzialità. Sarebbe infatti inutile e dannoso perpetrare o addirittura aumentare gli stanziamenti *sic stantibus rebus*. Che senso ha, infatti, fornire ulteriori risorse ad un'istituzione il cui corpo docente fatica a conquistare un accreditamento internazionale e dove gli studenti sono sempre meno preparati per affrontare il mondo del lavoro ad armi pari con i loro colleghi europei? nelle facoltà si è passati in 8 anni da circa 2.500 corsi di laurea e di diploma ad oltre 5.500 corsi di primo e secondo livello (per non parlare delle borse di dottorato erogate in ambiti disciplinari senza alcun valore scientifico), dall'altra parte, quella dei fruitori, il 20 per cento degli studenti lascia dopo il primo anno, mentre solo il 50 per cento degli immatricolati completa il ciclo di studi. Tutto ciò è avvenuto in assenza e ben prima dei famigerati tagli di Tremonti!

In quest'Aula il Partito Democratico ha recentemente accusato, a torto, la maggioranza e il Governo di aver dimenticato i giovani. Le novità introdotte dalla riforma dell'università proposta dal ministro Gelmini hanno però un valore simbolico altamente significativo: tali provvedimenti, integrati dai contributi provenienti dal dibattito in Commissione, che non tradiscono e piuttosto sottolineano il carattere riformatore del disegno di legge, indicano quantomeno una strada rispetto alla quale non si torna indietro e dalla quale ci auguriamo possano trarre vantaggio università virtuose, studenti e professori meritevoli. E allora, se vogliamo trovare il senso profondo di questo articolato provvedimento, lo rintracciamo forse nel convinto tentativo di riavvicinare finalmente l'università alla realtà. Le nuove generazioni, gli studenti che abbandonano prematuramente i corsi di laurea, e tutti quei laureati che non riescono a trovare un lavoro coerente al proprio investimento formativo chiedono all'università italiana una sola cosa: percorsi didattici spendibili nel mondo del lavoro. In altre parole, azzerare il distacco fra l'insegnamento universitario e la società reale. Lei, signora ministro Gelmini, ha meritevolmente seguito questa impostazione e nel farlo ha scelto di coinvolgere appieno il Parlamento, evitando lo strumento del decreto; ciò non toglie, tuttavia, che la materia non rechi elementi di urgenza e indifferibilità. In questo senso, desidero unirmi all'auspicio che il presente disegno di legge ottenga pronta approvazione nei due rami del Parlamento, trovando il voto favorevole di una maggioranza più ampia.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch'io partecipo per qualche breve minuto alla discussione generale, innanzitutto per complimentarmi con il Governo Berlusconi, con la signora ministro Gelmini, con il sottosegretario Viceconte

del corpo universitario, andando a toccare una delle criticità fondamentali nel sistema Italia. Mi complimento anche con il relatore,

e riguarda ormai un terzo dei corsi di laurea. A livello nazionale sono infatti a numero chiuso i corsi di medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie, architettura e scienze della formazione. Ogni anno in Italia tentano di accedere, soltanto nell'area sanitaria, circa 300.000 ragazzi, avendo a disposizione - come nell'anno accademico 2010‑2011 - per medicina e chirurgia solo 8.775 posti, per odontoiatria 789 e per veterinaria Diversi TAR, nel corso degli anni, hanno dato ragione agli studenti esclusi dalle facoltà di medicina e odontoiatria: solo per l'anno accademico 2009-2010 sono stati circa 7.000 i ricorsi pendenti. I criteri della selezione sono basati su un test articolato in 80 quiz formulati su cinque opzioni di risposta su argomenti di logica, cultura generale, biologia, chimica e fisica. La criticità di questo sistema risiede nel fatto che da questi 80 quiz emerge un grandissimo fattore di casualità e, al massimo, criteri di tipo nozionistico. Un'altra criticità risiede nella determinazione del numero dei posti, che viene effettuata con un calcolo presuntivo, soltanto su base nazionale, di quello che dovrebbe essere il fabbisogno del mercato lavorativo. In realtà questo criterio non ha alcun valore nell'ambito di una logica europea e non è predittivo nell'ambito di diverse annualità,

quella di «promuovere tutte le iniziative appropriate a risolvere, attraverso una nuova regolamentazione della legge, le incongruenze tra diritto allo studio e test d'ingresso, (...) rimodulando le prove d'ingresso e valutando in maniera approfondita le qualità e le capacità

circa il 20 per cento degli iscritti alle facoltà di medicina non arriva alla laurea. Allora, forse sarebbero opportuni margini più ampi al momento dell'ammissione, prevedendo degli *step* reali e concreti di maggior selettività

*(PD)*. Signora Presidente, caro Ministro, signor relatore, signor presidente Possa,

ora in Aula ad affrontare il disegno di legge che si è riproposto - o si era riproposto - di costituire un progetto parlamentare. Il lavoro svolto è stato proficuo e importante. Signor Ministro, mi consenta dunque in questo momento di approfondire alcune considerazioni e rilievi critici che a più riprese, in Parlamento e nella discussione pubblica, ho già avuto modo di svolgere e di rivolgerle. Questo disegno di legge è stato definito una riforma dell'università e questa riforma è stata definita mesi fa una opportunità storica.

alcuni motivi legati al malfunzionamento della nostra università; sono stati addotti addotti motivi legati al corrompimento, se non addirittura ad alcuni episodi di corruzione. Ciò che rende necessaria la riforma della nostra università non è legato

La radice principale che rende necessaria la riforma dell'università europea, e quindi anche di quella italiana,

poi la radicale trasformazione dell'organizzazione dei saperi, soprattutto nella frontiera delle conoscenze. L'esigenza di una riforma dell'università era stata posta dai grandi sommovimenti sociali che avevano preso

connesse al passato della nostra società. Non possiamo non rilevare che è finito il mondo all'interno del quale la grande riforma, più volte designata sotto il nome

Questa opportunità storica, signora Ministro, signor relatore, si è rivelata un'opportunità mancata. Questo disegno di legge, infatti, è collegato ad un enorme taglio, e di fatto - mi scusi, signora Ministro, la provocazione - siamo passati dalla riforma Gelmini ad una riforma Tremonti: è prevalso

da lei proclamati e, come lei sa, da me in larga parte condivisi all'inizio del suo Ministero. In sostanza, si tratta di un taglio su più fronti, una significativa riduzione di investimenti, dunque un taglio economico-finanziario che colpisce quattro grandi risorse della nostra università. Innanzitutto, un taglio un taglio di 1.300 milioni di euro per il 2011: ciò, come affermano gli stessi rettori e come a lei stessa, Ministro, i rettori hanno comunicato, corrisponderà di fatto al fallimento della maggior parte degli atenei pubblici italiani.

del nostro Paese, che non può essere umiliata o tagliata in questo modo, non solo per il loro interesse e per la loro dignità, ma anche per l'interesse culturale ed economico del nostro Paese e della nostra università. Questa riforma colpisce poi gli studenti, il diritto allo studio, il loro *welfare* e, soprattutto, la loro mobilità. Nulla è contenuto nel combinato disposto riforma Gelmini-riforma Tremonti che sia volto a valorizzare nel merito la mobilità, il *welfare*, il diritto allo studio. E questo è un discorso di meritocrazia, non è semplicemente una questione di economia.

abbiamo ascoltato in audizione - dalla Confindustria, oltre che dagli attori del mondo accademico, sono contraddetti proprio dal disegno di legge C'è da domandarsi perché tanto consenso sui principi ispiratori abbia prodotto un disegno di legge che li contraddice radicalmente. I principi ispiratori sono quattro: l'autonomia dei singoli atenei, vincolata invece in questo disegno di legge da decine di norme centralistiche; la promozione della responsabilità, impedita di fatto dalla risibile autonomia; la valutazione dei risultati della ricerca e della didattica dei singoli atenei (ma senza autonomia e responsabilità non si saprà che cosa valutare, soprattutto con un'Agenzia della valutazione (ANVUR) privata di risorse e di competenze adeguate); infine, il Il quarto principio, che è la bandiera della sua filosofia, da oggi sarà soltanto un proclama vuoto di contenuti, per due ragioni: senza sostegno alla qualità della formazione e della ricerca il merito non potrà emergere, e senza sostegno al diritto allo studio non potrà emergere il merito degli studenti meno abbienti. Questo è un fallimento grave, visto che la ricerca e la formazione superiore sono condizioni indispensabili per uscire dalla gravissima che stiamo vivendo e per mantenere ancorato il nostro Paese all'Europa, attraverso il conseguimento degli obiettivi concordati a Lisbona 11 anni fa. La preoccupazione mia e nostra è grande. Per questo abbiamo contribuito a migliorare con emendamenti il testo in esame, ma anche per questo motivo la nostra preoccupazione per l'università, per la mancata centralità dei giovani e degli studenti si traduce in una grave preoccupazione per il futuro sociale ed anche economico del Paese.

il disegno di legge sulla riforma universitaria arriva oggi all'attenzione dell'Assemblea dopo mesi d'intenso, proficuo lavoro nella Commissione 7a. La necessità di un riordino del sistema si era posta sin dall'inizio della legislatura, allorquando fu emanato il decreto‑legge n. 180 del 2008, che introduceva alcuni interventi urgenti sulle commissioni di concorso, sul reclutamento, sulla valutazione dei risultati, sulla premialità e sul diritto allo studio. In tale direzione si colloca il disegno di legge n. 1905, che ha, però, l'obiettivo più ambizioso di innovare la *governance* degli atenei e di ridisegnare l'intero settore all'insegna dell'efficienza e della valorizzazione dei meritevoli. L'università rappresenta, infatti, il luogo alto del sapere, dove le conoscenze, attraverso la libera circolazione delle idee, producono effetti non sempre tangibili e immediati, ma di sicuro impatto nel medio e lungo termine. Un Paese che non abbia come obiettivo la promozione del talento e delle idee, la cui fucina è senz'altro l'università, non può pensare di reggere alle pressioni della modernità e alla velocità del divenire. L'esame del provvedimento governativo ha rappresentato un'importante occasione proprio per confrontarsi, non tanto e non solo in ambito parlamentare, quanto soprattutto con gli operatori del settore sulla finalità di una, per noi, importante riforma. Delineare gli scenari possibili già nel breve periodo è stato dunque avvertito come una priorità, nella consapevolezza di dover creare una salda cerniera tra passato e futuro, senza però dimenticare le positive esperienze già maturate. Gli atenei, del resto, sono organismi di alta cultura, cui la Costituzione riserva un ruolo peculiare proprio in virtù del loro essere motori del sapere. Il testo governativo giunto in Commissione era, per la verità, a mio avviso, non del tutto esaustivo sul piano delle correzioni da apportare al sistema, nell'ottica di evitare distonie e sovrapposizioni di competenze; il lavoro svolto è stato dunque molto fruttuoso e approfondito, per limare quell'eccesso di prescrittivismo che caratterizzava il provvedimento nella sua formulazione originaria e salvaguardare in maniera idonea l'autonomia universitaria. L'attività emendativa ha consentito quindi di portare in Assemblea un disegno di legge per certi versi semplificato, per altri arricchito rispetto ad alcune carenze riscontrate nella proposta iniziale dell'Esecutivo, con riferimento agli stessi principi ispiratori di cui all'articolo 1. In questo senso, gli emendamenti da me presentati in Commissione avevano la finalità di modificare il testo a partire dalla sua formulazione letterale, fino ad inserire precisazioni doverose in un'ottica, penso, di maggiore chiarezza. Molte proposte sono state, in verità, recepite dallo stesso relatore, mentre altre, spero, potranno trovare un ulteriore terreno di confronto in questa fase. Senza dubbio alcuno il cuore della riforma sta nel mutamento della *governance*, che gli atenei sono tenuti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto disposto dall'articolo 2. In questo quadro, l'obiettivo di migliorare la competitività si persegue anche attraverso accordi di programma tra singole strutture e Ministero, tenendo conto dello sviluppo regionale. Si vuole favorire, cioè, un innalzamento della qualità senza un livellamento generalizzato, a partire, però, dalle reali condizioni di contesto. La misura mira, dunque, a promuovere iniziative individuali, oppure di gruppi di atenei, su base regionale e soprattutto a sostenere quelli svantaggiati, fissando pertanto parametri diversificati. La modifica è stata il frutto di un emendamento a mia firma, unitamente a quella del senatore Firrarello, che ha raccolto il consenso della Commissione, nell'ottica di innescare sinergie virtuose. L'idea di fondo sottesa al testo è di fissare linee generali di intervento, che la Commissione ha tuttavia talvolta limato per rispettare l'autonomia universitaria, in modo che il sistema accademico si ammoderni e superi le attuali storture, attraverso maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione. I rapporti tra gli organi di governo devono quindi essere ridefiniti, stabilendo con certezza compiti e durata degli incarichi (anche per evitare inutili sovrapposizioni) e valorizzando adeguatamente la componente studentesca, parte integrante della vita di ateneo. Non è un caso che le modifiche più significative siano state apportate proprio agli organi di vertice, consiglio di amministrazione e senato accademico: il primo ha funzioni più marcatamene esecutive, oltre che disciplinari, e con un'innovazione decisiva rispetto alla legislazione in vigore; il secondo invece ha un ruolo di proposta e programmazione, e può per la prima volta sfiduciare il rettore con qualificate maggioranze. Altra novità di rilievo concerne la fissazione di un numero minimo di componenti il consiglio di amministrazione esterni all'ateneo, proporzionalmente al totale dei membri, in modo da non paralizzarne le decisioni; ciò dovrebbe stimolare maggiormente l'apertura dell'università all'esterno e invogliare gli scambi reciproci con il mondo delle professioni e del lavoro. Il disegno di legge è permeato peraltro di misure volte a valutare la qualità della didattica e della ricerca, compito affidato a diversi soggetti a vario titolo operanti nell'ateneo come, ad esempio, l'istituenda commissione paritetica docenti-studenti. Per dare concreta attuazione alle finalità del testo e all'insegna di un'effettiva trasparenza, ho condiviso la modifica volta a sostituire il codice etico con quello deontologico, più correttamente attinente all'esercizio della professione. È pur vero che una parte consistente della riforma sarà affidata a decreti legislativi, con riguardo alla valorizzazione della qualità, dell'efficienza, della figura del ricercatore, alla contabilità, alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei

Gli articoli da 6 a 10 introducono norme direttamente applicabili e hanno riequilibrato l'impegno dei professori e ricercatori in rapporto alle attività di didattica e di ricerca nei due regimi del tempo pieno e di quello definito. Come ricordato anche dal relatore, è stata eliminata la certificazione delle 1.500 ore di ricerca, che ora vale solo figurativamente e per la rendicontazione dei progetti di ricerca. Il provvedimento sperimenta poi una combinazione diversa per la selezione del personale docente, tentando di porre finalmente termine alle cattive pratiche conosciute fino ad ora. Sul punto, già il decreto-legge n. 180 del 2008 aveva recato innovazioni relativamente alle commissioni di concorso, ma il testo all'esame si spinge oltre: esso istituisce, anzitutto, un'abilitazione nazionale quadriennale distinta per settori concorsuali che raggruppano più settori scientifico-disciplinari per la fascia di accesso alla professione; per i possessori dell'abilitazione è prevista in seguito una fase locale, regolata però da criteri indicati dalla legge, ancora una volta con l'obiettivo di ridurre la discrezionalità e di stringere la connessione tra autonomia di scelta e responsabilità. Con specifico riguardo agli attuali ricercatori a tempo indeterminato, ho rilevato criticamente l'assenza nel testo governativo di una normativa transitoria che consentisse di inquadrare tali figure nel nuovo disegno legislativo, considerato che vi era una pesante discriminazione ai loro danni in termini di prospettive di carriera. Ho pienamente appoggiato, perciò, la modifica al testo nella parte in cui dispone che anche i ricercatori a tempo indeterminato - e non solo quelli a tempo determinato - che conseguano l'abilitazione da professore associato possono essere chiamati direttamente dagli atenei, secondo l'articolo 18, comma 6. Tuttavia, per il ricercatore a tempo determinato, di cui al medesimo articolo 18, avrei preferito che la maggiorazione del 30 per cento del trattamento economico fosse riservata ai titolari di contratti rinnovati, atteso che la gratificazione economica deve seguire una valutazione dell'operato già svolto.

che la si possa considerare come un gioiello che finalmente acquisiamo nel nostro ordinamento, se prima non eliminiamo alcuni cancri evidenti, terribilmente evidenti e terribilmente gravosi su un'economia, quella italiana, che certamente è in difficoltà. Le riporto due esempi che ho vissuto dove svolgo la mia attività editoriale. Parliamo di Campobasso, la più piccola delle Regioni italiane ha istituito la facoltà di medicina, perché bisognava sistemare qualcuno. Lo dicono tutti.

Quindi, che necessità c'era di quella facoltà? Sta là dove c'è un sempiterno rettore di nome Cannata, che ha scoperto una novità assoluta: se termina il periodo - consentito anche dalla sua riforma - si trasferirà a Cassino: cosicché di Cannata ce n'è sempre uno. Ma quel che è più grave è che a Cassino, dove va, i due terzi dei docenti non hanno che sei, sette, al massimo otto studenti. Poi, a tutto questo aggiungiamo che il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione è privo anche di un qualsiasi diploma: ha fatto solo la terza media,

sgombriamo subito il campo da un equivoco: questo provvedimento non è una riforma innovativa, ambiziosa del sistema universitario. Questo provvedimento è assolutamente inadeguato a ridefinirre la configurazione della ricerca e dell'università nell'epoca dell'economia della conoscenza e della globalizzazione. Nonostante un serio lavoro emendativo, che ha fatto dire al relatore Valditara, giustamente, che il Parlamento non è stato un mero portavoce del Governo, la nostra contrarietà rimane netta, perché l'impianto di fondo non è stato scalfito. Ci troviamo di fronte, infatti, ad un modo di intendere il lavoro intellettuale che, come nel caso del provvedimento sugli enti lirici, appare improntato ad una seria incomprensione, sottovalutazione o, peggio ancora, a fastidio. La sottolineatura in alcuni momenti quasi furiosa, degli sprechi, in realtà copre una lontananza rispetto alla dignità del lavoro intellettuale, non utile immediatamente. Copre la consistentissima riduzione di risorse per l'università e la ricerca. Non che non ci sia bisogno di interventi per ridurre sprechi e improduttività, ma qui ciò che manca è un progetto in grado di chiamare a raccolta le maggiori energie dell'università e del Paese perché l'università e la ricerca siano un volano fondamentale dello sviluppo del Paese e della sua ripresa. Invece l'approccio verso chi vive e lavora all'università è punitivo. Il Governo e il ministro Gelmini si presentano come castigamatti che dicono: la ricreazione è finita. È da mesi, signora Ministro, che sentiamo ripetere, anche con una certa petulanza e dagli ambienti più diversi, le parole «autonomia», «responsabilità» e «meritocrazia». Figuriamoci: parole sante, ma sinceramente una presa in giro, se non si portano a soluzione tre grandi questioni prioritarie per un vero cambiamento dell'università: reale investimento su ricerca e università, numero di laureati in relazione agli iscritti e reale meritocrazia. Sul primo aspetto è chiara l'alternativa: o si investe o non si investe. L'Italia ha fatto di più: non investe e taglia, nonostante l'Italia occupi l'ultimo posto, tra i Paesi OCSE, per risorse all'università. il ministro Tremonti ha dettato il suo modello di risanamento e un modello di sviluppo che non prevedono la ricerca. E lei, signora Ministro, ha detto: va bene. Anzi, ha perfino pregato di non sollevare la questione delle risorse per non rallentare l'*iter* del provvedimento. Nell'articolo 1, nel definire il ruolo dell'università non vi era cenno a quello di luogo prioritario della ricerca e di elaborazione, riducendosi la missione dell'università a solo luogo di circolazione delle idee. In Commissione lo abbiamo modificato, maggioranza e opposizione, ma resta un impianto che non concepisce la grande ricerca e l'alta cultura come ingredienti fondamentali anche per l'innovazione tecnologica. È l'errore questo. In America le università questo punti di riferimento internazionale. I privati ne hanno un ritorno positivo anche per l'innovazione tecnologica e per questo investono molto. Da noi si fa l'opposto: si riduce la ricerca teorica, quella non spendibile a breve, solo sul breve; e così, un certo pragmatismo sbrigativo, anche il mondo economico: non solo non investe sull'università, ma rischia di piegare quest'ultima a fare da supporto a innovazioni non in grado di competere nel mondo. Così si prefigura la via del declino. Così come ha detto Israel in un bellissimo articolo apparso su un quotidiano romano, Obama identifica la forza dell'America con la forza della ricerca e per questo, nonostante la crisi, la ricerca rimane una scelta fondamentale. E sulla meritocrazia, sembra di udire Musil quando, ne "L'uomo senza qualità", faceva rimbombare le sue pagine "Grande riforma! Grande riforma!". Qui, invece, ad ogni piè sospinto sembra riecheggiare «Meritocrazia! Meritocrazia!». Ma come si fa a parlare di meritocrazia quando non la si lega alla produzione dei docenti,

Una vera riforma è quella che ricomincia ad investire sull'università come luogo di alta cultura, di ricerca di alto livello e di insegnamento a giovani che meritano, anche quando il reddito delle loro famiglie non è in grado di sostenere il loro valore.

tagli invece di investimenti, come sarebbe necessario: questa è la sintesi dell'operazione che il Governo sta compiendo e che mette in serie difficoltà il nostro sistema universitario pubblico. Mentre altri Paesi europei hanno risposto alla crisi, aumentando gli investimenti in formazione e ricerca, il ministro Tremonti ha pensato bene, ancora prima della crisi nel 2008, di operare un bel taglio di un miliardo e mezzo circa. Evidentemente, ha ritenuto che l'università dovesse essere fra i soggetti da punire. Eppure, in Italia si spende per l'università molto meno delle medie europea e OCSE e siamo nelle ultime posizioni per percentuale di laureati. C'è da intervenire e da cambiare? Certo. E noi siamo stati i primi a presentare le nostre proposte anche in questa legislatura, con riforme vere, cioé accompagnate da investimenti. Senza risorse, signora Ministro, nessun riforma potrà mai fare il miracolo di salvare e rilanciare la nostra università. il testo del Governo ha subito molti cambiamenti in positivo Commissione , grazie soprattutto a un'attività responsabile di tutta la Commissione e alla disponibilità del relatore, che voglio ringraziare. Molti nostri emendamenti migliorativi sono stati accolti e ora possiamo lavorare su un testo meno centralistico, meno burocratico e, mi consenta, meno ottuso. Ma ancora non ci siamo. Restano criticità importanti, che sono state richiamate dai colleghi che mi hanno preceduto. La prima e più importante riguarda i giovani, i giovani, che risultano essere i più penalizzati da questo provvedimento: penalizzati nel diritto allo studio, quello vero, che promuove la mobilità sociale e premia gli studenti meritevoli, nonché privi di mezzi, come recita la nostra Costituzione. il merito, signora Ministro, previsto all'articolo 4, è una vera e semplice finzione, priva di efficacia, non disponendo di una seria e certa copertura finanziaria, come anche il relatore ha riconosciuto nella sua relazione. In secondo luogo, vengono penalizzati i giovani che desiderano intraprendere la carriera accademica. Su questo, già era poco convincente il testo originario del Governo, che prevedeva la figura del ricercatore a tempo determinato per un triennio rinnovabile, prima della possibilità di assunzione come docente associato. Poco convincente soprattutto per il fatto che non viene previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. E, senza un accompagnamento oculato con le risorse necessarie all'assunzione, si creano soltanto illusioni e frustrazioni nei giovani, cosa che non vogliamo. Ma l'emendamento all'articolo 18 presentato per l'Aula dal relatore peggiora ulteriormente a nostro avviso, la condizione dei giovani studiosi perché allunga indiscriminatamente il periodo di incertezza e di precarietà. Misure positive sono state introdotte in Commissione riguardo ai ricercatori a tempo indeterminato, anche per volontà nostra, perché sono stati accolti i nostri emendamenti, che invece in base al testo del Governo erano lasciati senza futuro. Nessuna delle nostre proposte è stata invece accolta per i ricercatori a tempo determinato, figure create dalla precedente legge Moratti. Mi auguro - e la disponibilità del relatore in questo senso ci conforta - che in Aula vengano approvate misure concrete che non chiudano la strada ai giovani ricercatori ricercatori più meritevoli, che vogliono essere giudicati in base al loro valore, ma anche avere serie, reali e vere opportunità di ricerca accademica. accademica. Colleghe e colleghi, un Paese che non si prende cura dei giovani e della loro intelligenza è un Paese destinato al declino. E questo purtroppo è il rischio che corriamo come Paese. Noi questo non vogliamo accettarlo, non lo accettiamo, e faremo di tutto per cambiare, con grande senso di responsabilità,

Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla riforma universitaria rappresenta, io credo, l'acquisita consapevolezza dell'importanza che il sistema università riveste nel nostro Paese, della sua rilevanza strategica per la ripresa dello sviluppo economico, civile e culturale della società. Per la prima volta, dopo molto tempo, il legislatore interviene con una riforma a 360 gradi del complesso ordinamento universitario. Sono note le difficoltà e le contraddizioni che da decenni affliggono il sistema universitario e sono altresì note le esperienze di non adeguata gestione che hanno contraddistinto spesso l'utilizzo dell'autonomia da parte di numerosi atenei. Ecco perché l'ampia articolazione del disegno di legge costituisce una traccia importante, dando luogo a un modello organizzativo che si sforza di ribadire il rispetto dell'autonomia universitaria, ma rimarcando le responsabilità che derivano da tale libertà. Tutto l'impianto normativo s'incentra su una maggiore autonomia delle università e su un sistema di valutazione che vuole garantire sempre maggiore qualità della didattica e della ricerca universitaria. È evidente che l'autonomia delle università è un valore soltanto nella misura in cui è usata bene e, se presenta delle falle, è necessario accompagnarla con criteri e regole adeguate. Così come è necessario che le università elaborino programmi e progetti e che siano valutate e finanziate a seconda di come li realizzano. Ed è per questo che la valutazione deve essere accompagnata da un'azione premiale o sanzionatoria, in base ai risultati ottenuti dagli atenei nell'assegnazione di una quota delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università. D'altronde, va rilevato che lo stesso corpo accademico ha finalmente compreso che bisognava dare un taglio alle errate politiche universitarie di spreco e che l'offerta universitaria doveva adeguarsi alle reali esigenze del Paese, in particolare a quelle legate allo sviluppo occupazionale, volano necessario per la crescita di fiducia delle nuove generazioni nel futuro. Non scenderò nei dettagli della legge, che è stata già esaurientemente illustrata, ma mi soffermerò brevemente su alcuni aspetti che denotano il coraggio di questa riforma universitaria. A cominciare dalla *governance* degli atenei, che, definendo senza ambiguità compiti e ruoli degli organismi e separando la gestione politica da quella amministrativa, garantirà maggiore capacità decisionale, evitando mediazioni e tempi biblici. Oggi, infatti, assistiamo a un'inutile sovrapposizione di funzioni tra il consiglio di amministrazione e il senato accademico, che spesso ha reso particolarmente difficile la gestione degli atenei. Rivoluzionaria appare inoltre la presenza nel consiglio di amministrazione di soggetti esterni ai ruoli dell'università, benché minima, per il timore che con l'apertura al mondo imprenditoriale si potesse verificare un condizionamento da parte del capitale e una contaminazione della ragione di essere dell'università, che deve essere quella di produrre sapere. Ma non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, soprattutto davanti all'esigenza che l'università dialoghi con le forze produttive per creare un ponte tra formazione e lavoro e per incentivare la ricerca, volano necessario alla crescita del Paese. Onorevoli colleghi, questa innovazione non viola né lede la libertà e l'indipendenza delle scelte accademiche, ma consentirà l'afflusso di maggiori risorse finanziarie il cui utilizzo rientrerà nella responsabilità degli organi dei singoli atenei che potranno consentire anche alla ricerca di base e alle discipline economicamente più deboli di riconquistare la loro dignità. È vero, come titolava qualche giornale, che con questa riorganizzazione del sistema universitario si vuole introdurre nei nostri atenei più rigore e più merito. L'attualità ci impone il rigore e allora non ci si può scandalizzare se si procede a una seria razionalizzazione. Quasi 300 sedi, migliaia di corsi di laurea con pochissimi iscritti, oltre 2.000 corsi di dottorato, sono cifre che indicano una deflagrazione del nostro sistema universitario, mentre sarebbe importante chiedere ad ogni ateneo di concentrarsi su quanto sa far meglio, con maggiore vantaggio per la collettività. Allo stesso modo è importante che il testo normativo preveda che le singole università, per far fronte a situazioni di dissesto economico, potranno fondersi o federarsi tra loro anche limitatamente a specifici settori di attività. Rigore, ma anche merito, che vede la sua più alta manifestazione nell'istituzione del fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca. È vero che, come ha sagacemente osservato qualcuno, con questa legge entra un po' di riforma

È vero che, come ha sagacemente osservato qualcuno, con questa legge entra un po' di riforma Brunetta nell'accademia, attraverso la valutazione triennale dei docenti necessaria a riconoscere gli scatti stipendiali e la possibilità per loro di far parte delle commissioni che selezionano i docenti e valutano i progetti di ricerca. Ma tutto sommato, come scrive Galli Della Loggia, almeno un premio Nobel e un docente fannullone ed assenteista non percepiranno più lo stesso stipendio. Credo che dobbiamo apprezzare l'enorme sforzo compiuto dai colleghi in Commissione istruzione, e in particolare dal senatore Valditara, che hanno apportato importanti miglioramenti al testo, come quello fondamentale per la vita delle università relativo alla ricerca, che a differenza della didattica, non può essere conteggiata, perché un vero ricercatore non smette mai di fare il suo lavoro, neanche per strada. Ed era ora che venisse cambiato anche il meccanismo di reclutamento. Che ci piaccia o no dobbiamo ammettere che lo schema dei concorsi locali ha consolidato baronie e danneggiato giovani capaci e competenti. Mentre la nuova procedura di selezione è più semplice, più trasparente e più rapida e per di più responsabilizza le singole università che saranno chiamate a rispondere delle scelte compiute in sede di valutazione. Dicono che il grande assente della riforma sia lo studente. Eppure il Governo con chiare e precise disposizioni ha voluto garantire il diritto allo studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, ma non tralasciando premi e incentivi al merito a prescindere dalle condizioni economiche. In conclusione, credo che il Governo e il Parlamento abbiano imboccato la strada giusta. E che il futuro, pur con qualche sacrificio, restituirà alle nostre università prestigio, rendendole allo stesso tempo moderne e maggiormente competitive; centri di produzione del sapere e scuole di formazione per i nostri giovani che saranno più maturi e maggiormente equipaggiati per il competitivo e selettivo mondo del lavoro.

Signor Presidente, colleghe e colleghi del Senato, signora Ministro, la maggioranza che oggi governa si era posta in origine obiettivi non troppo lontani da quelli della mia parte politica e sui quali una convergenza, magari parziale, avrebbe potuto essere costruita. La nostra università ha bisogno di profonda innovazione: nell'edificio selettivo ed elitario costruito nell'Ottocento per un corpo studentesco decuplicato nell'ultimo mezzo secolo ci sono solo posti in piedi. Il sistema è divenuto un luogo di parcheggio delle giovani generazioni anziché un'operosa officina di talenti. È afflitto da colpevoli sprechi, da insopportabili sistemi di padrinaggio, da non scusabili assenteismi; ha proliferato sedi e corsi, ha frammentato il sapere; ha spesso temuto le aperture internazionali e difeso il localismo. Va però anche ricordato che nell'ultimo decennio, con risorse costanti, ha raddoppiato il numero dei laureati, mantiene dignitosi livelli di ricerca nelle classifiche internazionali, produce laureati e dottori che ben competono nel mondo. Ci attendevano perciò una riforma con la erre maiuscola, tanto più in una fase strutturalmente favorevole come questa, nella quale ragioni sia demografiche, sia di saturazione non ci pongono di fronte al problema di espandere i numeri degli studenti (e quindi dei docenti), ma di selezionarli, incentivarli, formarli, qualificarli, impiegarli meglio senza perderne per strada la metà, come oggi accade. Ma al Governo è mancato il coraggio, e ci troviamo dì fronte, col disegno di legge in discussione, ad un pavido *bricolage*. Il provvedimento dà forse più risorse al sistema, riconoscendo la priorità della conoscenza nel cammino dello sviluppo? No, le riforme sono a costo zero, ma uno zero... nel negativo - mi perdonino i matematici - perché le risorse sono già state pesantemente tagliate e forse lo saranno anche in seguito. Si occupa di recuperare i finanziamenti privati, con un'intelligente politica fiscale? Giammai, non avesse ad offendersi il Ministro dell'economia! Dà sostanza ad una asserita ispirazione liberale, permettendo agli atenei di organizzarsi al meglio, seguendo la vocazione e l'opportunità? Non se ne parla nemmeno: si centralizza a tutto spiano. La sfiducia nell'università è tale che il piano strategico - che significa scienza e insegnamento - è approvato dal consiglio di amministrazione, organo tecnico-gestionale, anziché dal senato accademico, che è l'organo scientifico. Si dettano poi norme stringenti per l'organizzazione interna, precludendo agli atenei di articolarsi secondo logiche proprie. Incoraggia gli studenti che meritano? Solo a parole, con le medaglie di latta erogate dal Fondo per il merito, un salvadanaio senza denaro pubblico e con poca speranza di attrarre l'obolo privato. Si occupa del diritto allo studio? Ma quando mai: ci pensino le Regioni! Valuta il merito dei docenti, della ricerca, degli studenti? A parole, perché l'ANVUR, l'Agenzia di valutazione, è tuttora un guscio vuoto, ci sono piani (che si conoscano) per costituirne le capacità tecniche per fare il suo difficile mestiere. Si recluteranno i docenti migliori? C'è da essere scettici: si è congegnato un sistema doppio, dispendioso e poco efficiente. C'è un'abilitazione nazionale, senza limiti e tetti numerici, per ogni ambito disciplinare, i cui giudici - sorteggiati in una lista di "volontari" e che perciò può non selezionare i migliori giudici mentre sicuramente seleziona chi è interessato a sospingere i propri allievi - saranno sottoposti alla poco resistibile pressione di allungare la lista degli abilitati. C'è poi un "concorso" locale tra gli abilitati. Il primo sarà un filtro debole, il secondo una selezione influenzata dalle logiche locali. Viene affrontato il tema dello svecchiamento del corpo accademico? Non sembra proprio, e in più si pongono i ricercatori su un binario che, se non proprio morto, è moribondo, per assenza di finanziamenti. Signor Presidente, i principi sbandierati dalla maggioranza sono traditi dal disegno di legge: non si valorizza il merito senza risorse, non si valuta a parole senza costruire le capacità per farlo e l'Agenzia per la valutazione è un fantasma; non si coltiva la responsabilità centralizzando e togliendo autonomia. Il PD, che voterà convintamene contro questo disegno di legge, è pronto per una coraggiosa riforma, non per un *bricolage* dell'esistente. Due milioni di studenti, due milioni di famiglie, 100.000 persone che lavorano nelle università si attendono di più e di meglio. Gli auspici non sono positivi: il Presidente del Consiglio ha pensato bene di iniziare la settimana nella quale qui in Senato è approdata questa legge visitando un'università: ma non Harvard, non Oxford, non la Sorbona, non quella di Bologna, di Pisa o di Padova, bensì il *campus* di una neonata pseudouniversità telematica, l'unica che sia stata istituita (era ministro Letizia Moratti) nonostante il parere contrario del CUN.

Signor Presidente, ministro Gelmini, sottosegretario Viceconte, onorevoli colleghi, licenziando questo disegno di legge l'Aula del Senato porta un sostanziale e concreto contributo alla realizzazione di un preciso impegno che questa maggioranza assunse con gli elettori e contenuto tra le sette missioni per il futuro dell'Italia con riferimento a ricerca, università e cultura. Dopo la riforma della scuola, dunque, un importante altro passo in avanti verso l'attuazione del programma di governo che si compie nel segno di una reale svolta riformatrice con la precisa volontà di innovare in modo organico e strutturale un settore strategico per lo sviluppo del Paese, peraltro con un dibattito politico sull'argomento che ha occupato gli ultimi vent'anni, segnato anche da numerosi provvedimenti legislativi assai controversi. Sei mesi di lavoro in Commissione, sotto la sapiente regia del presidente Possa e con il responsabile impegno dei colleghi Asciutti e Valditara, che si è giovato di oltre 30 audizioni e di un serrato confronto cui anche l'opposizione ha fornito un apprezzabile contributo anche di tipo emendativo. Ortega y Gasset affermava: «L'università torni ad essere ciò che fu nella sua ora migliore: il principio motore della storia europea». e ricerca quali motori di sviluppo: credo sia questo il principio ispiratore della riforma in discussione ed è per questo che oggi la accogliamo con favore, apprezzando il lavoro sin qui svolto e auspicando che il dibattito possa produrre ulteriori miglioramenti ad un testo la cui *ratio* e il cui impianto sono apprezzabili e condivisibili, come è apprezzabile, signora Ministro, la sua scelta di presentare un disegno La storia delle riforme dell'università occuperebbe troppo tempo per essere ripercorsa, ma per comprendere l'inadeguatezza del sistema normativo sistema normativo vigente e dunque l'urgente necessità di riformarne il contenuto gioverà ricordare alcuni dati: nessuna delle 150 università italiane è tra le migliori 150 del mondo; 37 corsi di laurea hanno un solo studente iscritto; 327 facoltà non superano 15 iscritti; dal 1998 al 2006 il numero dei docenti è passato da 48.000 a 62.000 mentre è rimasto immodificato il numero degli studenti; abbiamo 94 università con ben 320 sedi distaccate situate non sempre in posizioni strategiche sul piano territoriale; abbiamo 170.000 materie insegnate rispetto ad una media europea di 90.000;

di nepotismo, di inefficienze e di sperperi di denaro pubblico che leggiamo non di rado negli occhi disillusi di tanti, tantissimi giovani capaci a cui è stato rubato il futuro. Di giovani talenti che trovano fortuna, successo e gloria molto spesso lontano dalla loro terra, di cui ci ricordiamo solo quando salgono agli onori della cronaca internazionale con riconoscimenti al loro impegno: ce ne ricordiamo quando, però, purtroppo, è troppo tardi e demagogicamente ci limitiamo a dissertare della fuga di cervelli, della genialità *made in Italy* più apprezzata all'estero che non in Patria, men che meno nel nostro Mezzogiorno, quel Mezzogiorno generoso tributario di tante intelligenze al villaggio globalizzato delle scienze e della ricerca. però, anche i numeri della crisi che ci spiegano le difficoltà antiche di un corpo accademico evoluto e prestigioso, quello virtuoso, quello che lavora, quello che produce e che fa onore all'Italia pur tra i mille guasti della burocrazia, quello che patisce i danni dell'autoreferenzialità, quello che rigetta e contrasta le logiche asfittiche di una tradizione - diciamo così - che si perpetua sulla spinta di interessi autoconservativi, di inconfessabili privilegi che soffocano il merito, di nepotismo che mortifica e avvilisce; insomma, una realtà che sembra scivolare verso il declino e nella quale i non pochi casi di eccellenza e di prestigio non sono più sufficienti a muovere efficacemente il volano della competitività che genera sviluppo e che usa il capitale umano quale fondamentale risorsa irrinunciabile per il progresso sociale, culturale ed economico dell'intera comunità. Fondo per il merito destinato a promuovere l'eccellenza tra gli studenti; premialità economiche per le università virtuose con la migliore produzione scientifica, didattica ed organizzativa; blocco delle assunzioni per le università con bilancio in rosso; procedura nazionale di reclutamento dei docenti con commissioni terze; norme per agevolare la soluzione del precariato per i ricercatori; rafforzamento delle procedure di valutazione scientifica attraverso l'ANVUR; semplificazione della *governance* interna con riequilibrio di funzioni tra senato accademico e consiglio di amministrazione: credo che con queste, che sono tra le principali innovazioni, la riforma che ci accingiamo ad approvare interpreti pragmaticamente le esigenze del cambiamento. E lo fa con coraggio e determinazione perché spinge il sistema universitario verso la cultura della buona amministrazione, della trasparenza e del riconoscimento del merito e delle eccellenze. Essa ricongiunge all'onore della spesa l'onere del risultato e coniuga l'autonomia decisionale ai principi del rigore, della trasparenza e della responsabilità. Siamo certi che il principio di responsabilità, pur lasciando impregiudicata l'autonomia degli organi decisori nelle scelte politiche,

per regolare l'orologio delle procedure concorsuali per finalità non proprio commendevoli, come ben ricordava Francesco Giavazzi qualche giorno fa dalle colonne del «Corriere della Sera», riferendosi ai «tempi eterni e alla corruzione dei concorsi che hanno indotto tanti giovani ad emigrare».

che vedono proiettato il nostro sistema universitario verso i migliori standard internazionali. Dal ministro Gelmini abbiamo ricevuto in questi mesi di lavoro la conferma della sua tenacia e della sua autorevolezza. Da esse traiamo la migliore garanzia che le risorse economiche destinate al comparto siano reperite quanto prima e nella misura adeguata alle esigenze di finanziamento che l'attuazione della riforma richiede, anche per un suo atterraggio morbido e completo in sede applicativa da parte degli atenei. Come pure auspico il suo impegno, signora Ministro, per il recupero degli scatti di anzianità per docenti e ricercatori a cui, sulla base di indici di produttività e di merito, gioverebbe un trattamento economico più adeguato ai sacrifici di una carriera lenta e complessa. Le saremo accanto, signora Ministro, anche nella doverosa sensibilizzazione del Governo e del Ministro dell'economia, affinché la necessaria dotazione economica consenta alla riforma che porta il suo nome di dispiegare i suoi indubbi positivi effetti. «Nessuno - neanche gli studenti - può negare la necessità di una riforma del sistema universitario», diceva qualche giorno fa da Trieste il presidente Napolitano, augurandosi che la discussione avviata in Senato portasse verso l'approvazione della riforma e spingendo tutti a fare autocritica. Il Presidente ha altresì detto: «Noi abbiamo avuto scelte discutibili e onerose, come la proliferazione delle sedi e dei corsi di laurea, fenomeni di inefficienze e disordine nella *governance* del nostro sistema universitario». Onorevoli colleghi, quello del Capo dello Stato suoni come un monito e sia l'occasione per consegnare al Paese, non solo una buona legge, ma anche l'immagine rinnovata di un Parlamento responsabile e capace di svolgere la sua funzione per il bene dell'intera comunità. Questa è un'occasione da non perdere!

empatici a dire esattamente ciò che avremmo voluto vedere in una vera riforma dell'università. Sono toni così poco ricchi di speranza perché lei ed io, all'inizio di questa legislatura, ci eravamo riproposte una vera riforma dell'università. Non avrei temuto nessun giudizio di inciucio se fossi riuscita a farmi capire dalla maggioranza, dal Ministro e perfino dal mio Gruppo, nel preparare una riforma che traguardasse le nostre persone. Una riforma universitaria deve valere tra 10-15 anni, ed è a quei giovani che dobbiamo pensare. Questa riforma non si interessa dei giovani, nemmeno di quelli che sono già all'università, perché quello che diciamo dei ricercatori è una presa in giro. Ciò che mi turba, di cui ho già sentito avvisaglie, che i colleghi della maggioranza che si erano espressi in Commissione con un certo tono e certi contenuti, in Aula li stanno cambiando. Capisco le esigenze dell'appartenere ad una maggioranza, ma amo molto il «sì sì, no no» anche in politica, e questa riforma, che rinvia continuamente ad altre sedi, ad altre norme, comincia subito con il negare la logica dell'autonomia. Una riforma vera avrebbe dovuto affidare all'autonomia dell'accademia la propria struttura e il proprio profilo. A quel punto la valutazione avrebbe fatto emergere una concorrenzialità che non c'è. Non c'è nemmeno, caro collega Calabrò, nelle rinnovate modalità del reclutamento. Credo che abbiate memoria, come me, del fatto che pochi mesi fa era stato detto in questa sede che avremmo fatto un reclutamento diverso, migliore e più trasparente. L'abbiamo alle spalle.

Per ora, sembra sia la sentina di tutte le corruzioni e incapacità. Ma se abbiamo ricercatori famosi nel mondo, se addirittura

in questo nostro disegno di legge potremmo avere dei rettori che fanno di mestiere il rettore, perché, se è vero che blocchiamo la possibilità che siano rinnovati nella propria università, possono però andare altrove.

Ho trovato un bellissimo testo, che credo in quest'Aula possa essere apprezzato da tutti, che recita: «L'università è l'istituzione che presidia la libertà del sapere e la tensione intellettuale alla verità, fornisce un contributo primario alla ricerca, garantisce i gradi più elevati della formazione, sostiene e dà metodo al confronto pubblico...». Il testo continua affermando che "appare cruciale quello che collega la necessità di crescita dell'autonomia anche finanziaria da parte delle università... e la necessità che lo studio e la carriera universitaria non siano rese impossibili a giovani capaci e meritevoli, privi però di adeguate risorse finanziarie". La parte del diritto allo studio è evanescente. All'inizio - pensate, colleghi, visto che conoscete la storia dell'università come me - le università non erano fatte per gli studi studi ma per gli studenti, i quali si tassavano e sceglievano un intellettuale che serviva loro per la formazione umana, intellettuale e civile. Questa riforma

realizzato. È pertanto con grande rammarico che rassegno a voi, che mi avete visto lavorare appassionatamente, la delusione per non poter votare una vera riforma. Grazie

che più volte ho rappresentato in quest'Aula e che riguarda i nostri giovani musicisti. L'apprendimento e l'insegnamento della musica siamo tutti d'accordo - devono essere incentivati sin dalla più giovane età. Se andasse in applicazione la legge n. 508 del 1999, che prevede

Ci sono molti colleghi senatori che sono anche colleghi accademici e ben sanno che l'università italiana in questo ultimo quarto di secolo è andata letteralmente alla deriva, per molti e molto gravi motivi: adotta pratiche di reclutamento familistiche e amorali, talora malavitose, che premiano, quando va bene, l'anzianità o i servizi resi più le capacità scientifiche e didattiche; non differenzia carriere e stipendi in relazione ai meriti ed ai risultati; ignora a tutti i livelli meritocrazia e standard di valutazione internazionalmente accreditati; moltiplica - lo abbiamo visto nei numeri - corsi dai nomi improbabili e dalle prospettive professionali assolutamente inconsistenti; non chiede agli studenti un alto livello di impegno e di studio e non offre loro una cultura e una formazione adeguate; per contro, impone tasse sempre più alte, vendendo in fondo quello che le rimane perché è garantito da un monopolio di legge che non avrebbe ragione di essere, ossia il monopolio del valore legale del titolo di studio, quello che quel pezzo di carta garantisce. Così facendo, si ripropone anche una sorta di selezione sulla ricchezza, che è il contrario dell'uguaglianza delle delle opportunità, che dovrebbe essere il fondamento di una società aperta. Il problema non è tanto, e non solo, l'assenza di risorse, ma un certo egualitarismo che ha ucciso il merito: quarant'anni di sbronza egualitarista hanno prodotto generazioni di somari che si sono anche riprodotti e sono anche andati in cattedra, e ne vediamo oggi i risultati. In questi anni abbiamo visto di tutto, ad esempio nel reclutamento, con la sanatoria conseguente alla riforma del 1980, che ha imbarcato una marea

che ha creato, con quei concorsi locali, incredibili idoneifici, mercati delle idoneità retti dai baroni che localmente cercavano di difendere e di blindare - in genere con successo - la posizione di spesso impresentabili candidati interni, indigeni. La contemporaneità di moltissimi concorsi locali ha favorito, del resto, ogni genere di trattative perverse tra le commissioni, con i casi limite, ben noti a tutti, di persone che potevano essere contemporaneamente giudicate da un commissario ed essere colleghi di quel commissario in un'altra commissione, che si svolgeva nello stesso momento in un altro ateneo. Abbiamo visto di tutto e forse anche di peggio dal punto di vista della didattica, con la moltiplicazione di corsi e insegnamenti, realizzata affinché pesassero di più i docenti che volevano ritagliarsi o valorizzare le proprie aree disciplinari, magari ristrette. Abbiamo assistito al riscorso oceanico all'istituto del professore a contratto: talvolta oltre la metà dei corsi di una facoltà erano tenuti da docenti scelti, senza concorso e senza controllo, dai soliti baroni, che in qualche modo favorivano i loro mediocri amici, quando non parenti, i quali si fregiavano - e si fregiano tuttora - del titolo di professore a contratto per trarne benefici nelle loro attività professionali. Abbiamo visto una concorrenza al ribasso, a tutti i livelli, tra insegnamenti, tra facoltà, tra università, basata sul fatto non di cercare l'eccellenza nella didattica e nella ricerca, ma al contrario di attrarre studenti nella misura maggiore possibile per poter acquisire importanza e finanziamenti (salvo poi liberarsi di quegli stessi studenti nel modo più rapido e indolore possibile, con esami

Si potrebbero aggiungere molte altre cose: sulla mancata differenziazione del triennio iniziale tra chi prosegue per il quinquennio e chi invece cerca una formazione professionalizzante; sull'inadeguatezza di molti dottorati di ricerca, spesso senza attività didattica e senza una seria tesi di dottorato, come richiesto negli altri Paesi; sull'esiguità dei trattamenti economici delle persone che fanno il dottorato di ricerca o che sono assegniste di ricerca e, per la verità, sullo stesso sistema dei crediti, che ha educato gli studenti all'idea che se un'attività non comporta l'acquisizione di crediti non vale niente. Posso organizzare un seminario nella mia facoltà con un premio Nobel ma, se non attribuisco un credito per la frequenza, so che non verrà nessuno: questo è il messaggio che abbiamo dato agli studenti.

acrobazie organizzative e burocratiche per far quadrare le varie ondate di norme che si susseguono sugli ordinamenti didattici del «3 più 2» introdotto dalla riforma del 1998. Con l'autonomia degli atenei il tasso di burocratizzazione invece di diminuire è aumentato, perché non è stato decentrato un bel niente, ma ogni sede locale ha prodotto ulteriori stratificazioni di richieste burocratiche, che sono andate a pesare su un corpo docente ormai

sia pure perfettibile in alcuni punti, credo incontri ampiamente questa esigenza. Ritengo che la riforma abbia il pregio di valorizzare il merito e di ricollegare l'autonomia e la responsabilità. L'autonomia senza la responsabilità ha generato spese senza controllo, burocrazia, scarse risorse per la ricerca, follie nell'offerta didattica. Ora il finanziamento pubblico sarà erogato sulla base della qualità della didattica e della ricerca, valutata in modo indipendente, secondo criteri internazionali. Le commissioni sorteggiate, formate da soli ordinari, e l'abilitazione nazionale, che si svolgerà sotto gli occhi di tutti e non in sedi dell'estrema periferia,

giovane ha solo la speranza di andare all'estero. Ebbene, credo che questa riforma possa restituire loro la speranza di poter restare, che possa consentire all'università italiana di concentrare le risorse nei punti di eccellenza che, in parte, ancora esistono e che si possono ricostruire e che la strategia di premiare l'eccellenza per moltiplicarla possa finalmente permettere la concorrenza virtuosa fra gli atenei basata su corsi eccellenti, su prospettive di lavoro, al posto di quella concorrenza al ribasso fatta di studi facili, di voti alti e di titoli inutili di cui si L'università facile, inclusiva, che fa sentire tutti dei piccoli premi Nobel, ha creato, in realtà, dei disadattati e lo sfascio dell'università, come quello della scuola, ha fatto sì che in questi anni sempre di più in Italia si sia preferito cercare l'affermazione sociale ed economica non con la cultura e la conoscenza, ma sfruttando le fortune di famiglie, le relazioni, le raccomandazioni, le *lobby* partitiche. È un mistero perché ancora oggi si possano preferire queste selezioni spurie, immorali e sconce a quelle basate sui meriti personali, sull'impegno e l'entusiasmo che ciascun ragazzo può mettere nel proprio studio e ciascuno studioso può mettere nella sua attività di ricerca. Abbiamo il dovere di restituire all'istruzione e alla ricerca la possibilità reale di aumentare le capacità intellettuali e professionali e, solo per questa via, di offrire a chi le merita nuove opportunità di lavoro e di innovazione. Questa riforma ha un grande merito. Il suo successo, certamente, dipenderà anche dal lavoro dell'Aula e poi dalla sua attuazione, dai regolamenti che ne seguiranno, ma dobbiamo e possiamo con questa riforma restituire ai giovani e alle imprese del nostro Paese la fiducia nel fatto che lo studio e la ricerca sono davvero in grado di trasferire loro conoscenze, attitudine ad affrontare i problemi, prospettive professionali, innovazione, progresso in una società che torni a far corrispondere il successo e le opportunità all'impegno, all'assunzione di responsabilità, al merito; esattamente quello che a troppi di loro e a troppi italiani ancora oggi è negato.

onorevoli colleghi, rubo un paio di minuti ai colleghi di Gruppo, molto più autorevoli di me in questa materia, per sottolineare alcuni aspetti della riforma, ma soprattutto per ribadire alcune nostre posizioni in tema di università. Dalla discussione in Aula, nell'opinione pubblica e nei *mass* *media* si evince l'importanza di questo argomento che non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma interessa l'intera comunità nazionale. L'istruzione, l'università e la ricerca sono infatti l'investimento fondamentale per lo sviluppo del Paese, sono il futuro dell'Italia. Lo ha ribadito recentemente il presidente quando ha detto: "Non riconoscere la priorità dell'alta formazione e della ricerca significa non avere senso del nostro futuro, non avere senso dell'identità e del ruolo della Nazione italiana". Da questa consapevolezza trae spunto l'elaborazione che il PD ha compiuto in maniera approfondita in questi mesi, sfociata poi in proposte per una riforma vera, di ampio respiro e lungimirante.

come molti nel centrodestra hanno fatto in questi mesi - arrivare a conclusioni semplicistiche, ad una demonizzazione dell'intero comparto. Stiamo parlando di un organismo malato che ha grandi potenzialità e che va curato e rigenerato nel segno della qualità dell'alta formazione e ricerca. Partendo da questi presupposti, ci si aspettava una riforma vera, che guardasse al futuro. il disegno di legge, anche se migliorato nel corso dell'esame in Commissione, non va in questa direzione. Ricordo come all'interno delle università italiane ci sia la consapevolezza della necessità di cambiare, di razionalizzare, di ottimizzare le risorse. Molti atenei stanno ragionando e programmando la propria offerta formativa in quest'ottica, cercando anche a livello territoriale importanti sinergie. Vorrei portare come esempio le due università della Regione Friuli-Venezia Giulia, Udine e Trieste, Grazie all'interno dell'area regionale, ricca di istituti di alta formazione e centri di ricerca di eccellenza; essendo il Friuli-Venezia Giulia una Regione di confine, ci sono pure interessanti progetti con università austriache e slovene per migliorare la qualità formativa e consentire una maggiore mobilità transfrontaliera ed internazionale agli studenti. È questo uno dei motivi per cui sarebbe necessario garantire maggiore autonomia ai singoli atenei per consentire loro un legame più forte con il proprio territorio e le sue specificità. Tralascio la questione della riduzione dei fondi, per soffermarmi sul tema dei giovani, di cui abbiamo ampiamente discusso anche in occasione della manovra finanziaria, perché, come Partito Democratico, siamo convinti che non si possa bruciare la grande risorsa rappresentata dalle nuove generazioni. Esse vengono sistematicamente sprecate; le nostre proposte sono all'insegna del ricambio generazionale, dallo sblocco del *turnover* al pensionamento a 65 anni e all'attivazione di nuovi posti. Per i ricercatori si prevedono percorsi rapidi e certi al fine di abolire il precariato intellettuale. Rispetto agli studenti va garantito il diritto allo studio, come previsto dalla Costituzione. L'università non deve essere ingiusta verso i giovani, ma deve rappresentare il motore della mobilità sociale. Un'ultima notazione, o meglio raccomandazione: nell'ambito della razionalizzazione non vorrei venissero soppressi i lettorati di lingua slovena presenti nelle università di Roma, Trieste e Udine, previsti dall'accordo culturale tra i Governi italiano e sloveno. Stante la situazione geopolitica ed il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi in diversi settori, essi andrebbero rafforzati, anche attraverso professori di ruolo. *(Applausi dal

signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, il provvedimento alla nostra attenzione attua una profonda e coraggiosa riforma del sistema universitario nazionale, incidendo su suoi snodi fondamentali, quali in particolare la struttura di *governance* delle università, le procedure di reclutamento del personale docente, lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, le modalità di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, l'incentivazione della qualità e dell'efficienza, la promozione della cultura del merito. Il relatore nella sua approfondita relazione di giovedì mattina ha ben messo in rilievo quanto sia articolato e complesso l'intervento che si intende attuare con questo provvedimento. La sua incisiva azione si esplicherà mediante molte decine di precise disposizioni, mediante quattro rilevanti deleghe legislative (da attuare entro 12 mesi), mediante l'emanazione di vari regolamenti, decreti ministeriali e decreti interministeriali, mediante l'adozione da parte delle università di importanti regolamenti di ateneo, le cui linee guida sono stabilite nel provvedimento. Saranno necessari uno o due anni almeno, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, perché tutte le decisioni in essa contenute siano effettivamente rese operative. Il provvedimento costituirà una salutare medicina per varie patologie che soprattutto in quest'ultimo periodo hanno afflitto le nostre università, quali perniciose derive corporative, un reclutamento del corpo docente non sufficientemente attento alla qualità, l'eccessiva moltiplicazione delle sedi, la finanza allegra. La limitatezza del tempo a disposizione su un provvedimento così complesso mi obbliga a concentrarmi solo su alcuni punti rilevanti. Un primo aspetto meritevole di attenzione è la nuova concezione del sistema universitario alla quale si ispira il disegno di legge. viene superato l'obiettivo di un sistema universitario nazionale distribuito sul territorio in modo da realizzare la massima omogeneità per quantità e qualità della offerta formativa, obiettivo che è stato storicamente prevalente negli ultimi decenni, giustificato da comprensibili istanze di egualitarismo delle opportunità di studio, dalla gravemente insufficiente disponibilità di residenze studentesche e dalla volontà di riscatto del Mezzogiorno; obiettivo che è stato anche sostenuto in varie Regioni in funzione di specifiche politiche di sviluppo del sistema produttivo. Ad attuare tale cambiamento di politica universitaria sarà l'introduzione, prevista dal provvedimento, di

Le università che si dimostreranno più virtuose potranno così disporre di maggiori risorse, che consentiranno ad esse di diventare ancora più virtuose. In base alla disposizione del comma 2 dell'articolo 1, queste università virtuose potranno anche sperimentare (con l'accordo del MIUR) modelli organizzativi e funzionali diversi da quelli prescritti in via generale nel provvedimento. Obiettivo fondamentale del provvedimento è il miglioramento della qualità dell'attività del personale docente. Per il personale docente già in servizio tale miglioramento verrà ottenuto mediante periodiche valutazioni dell'attività, che se positive avranno vari effetti premiali. Al riguardo, la scienza del *management* è concorde nel ritenere sempre positiva l'azione di controllo della prestazione, purché i criteri di valutazione e le conseguenze premiali o punitive della valutazione siano *ex ante* chiare

Per l'università italiana si tratta di una innovazione molto importante. Basti pensare che a tutt'oggi, superato il periodo di straordinariato, il professore ordinario non è soggetto ad alcun tipo di valutazione. In generale, saranno le singole università ad avere competenza esclusiva circa la valutazione dell'attività di un professore o di un ricercatore nelle sue due espressioni della ricerca e della didattica e, a questo fine, definiranno nei propri statuti gli organi incaricati delle valutazioni e le relative procedure. Per tale nuovo compito, il provvedimento prevede, all'articolo 5, comma 3, lettera *e)*), un potenziamento dei sistemi di autovalutazione delle università, basato anche sugli attuali nuclei di valutazione. Il singolo docente o ricercatore verrà sottoposto a due differenti valutazioni periodiche personali. Ciascuna valutazione sarà a due livelli, positiva o negativa. La prima valutazione periodica personale è quella disposta dal comma 5 dell'articolo 6 Il testo del provvedimento non precisa esplicitamente la periodicità di questa valutazione (anche se forse sarebbe opportuno che lo facesse); a buon senso, dovrebbe trattarsi di una periodicità annuale. Per l'attività di ricerca ci si atterrà ai criteri oggettivi di verifica dei risultati stabiliti dall'ANVUR, utilizzando (presumibilmente) le informazioni contenute nella banca dati recentemente istituita contenente i dati relativi alle pubblicazioni dei professori e dei ricercatori. Per l'attività didattica ci si riferirà alle modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti definite nei regolamenti d'ateneo. In caso di valutazione negativa i professori e i ricercatori saranno esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. La seconda valutazione periodica personale è quella disposta dal comma 12 dell'articolo 6. In base a tale comma i professori e i ricercatori sono tenuti ad allegare alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale (ora triennale) una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio. Tale relazione costituirà la base per la decisione dell'attribuzione (o non attribuzione) dello scatto stipendiale triennale, decisione che sarà presa dalle singole università secondo quanto disposto dai regolamenti di ateneo. Sarebbe opportuna una disposizione che minimizzasse il rischio di valutazioni disomogenee tra le università: sarebbe poco accettabile che professori di diverse università, ma ugualmente efficienti in base alla loro relazione triennale, avessero trattamenti diversi anche in termini di scatto stipendiale. In ogni caso, occorrerà fare molta attenzione a non ledere in queste valutazioni personali i fondamentali diritti di libertà di insegnamento e di ricerca che sono costituzionalmente garantiti per chi opera nell'università. L'attività dei professori (e ricercatori) verrà sottoposta anche ad altre valutazioni. All'articolo 5, comma 2, è prevista, per potenziare la capacità di autovalutazione dell'università, l'istituzione in ciascun dipartimento o facoltà di una commissione paritetica docenti-studenti, che avrà tra l'altro il compito del monitoraggio della qualità della didattica.

interne. Il comma 1 dell'articolo 1, che ha come sottotitolo «Princìpi ispiratori della riforma», ribadisce molto opportunamente che le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione e luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza e, richiamandosi al modello humboldtiano di università, sottolinea sottolinea che le università «operano combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». L'argomento merita un approfondimento. Ricercare ed insegnare sono due azioni molto diverse, richiedono modalità attuative, culture, attenzioni, linguaggi, forme di comunicazione tra di loro assai diverse, spesso divergenti. Questo stretto connubio tra ricerca e didattica ha caratterizzato con grande successo l'università di *élite*, che per tanti decenni è stata l'espressione dell'alta formazione nel mondo occidentale. Tuttavia, tale esigenza non è più così indispensabile, a mio avviso, per un'università divenuta di massa. In Italia accede attualmente all'università un'imponente massa di giovani, una frazione considerevole della popolazione giovanile, oltre il 40 per cento. Nel 2007 i laureati in Italia sono stati circa 300.000, di cui 51.040

L'Italia è ormai diventato uno dei Paesi al mondo che sforna annualmente più laureati. Alla grande maggioranza di questi giovani occorre fornire nelle varie discipline gli elementi fondamentali necessari ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, elementi che sono ormai molto distanti dal fronte delle conoscenze. A tale fronte verranno fatti accedere con studi impegnativi solo i pochi che vogliono intraprendere con il dottorato di ricerca

si sono progressivamente consolidati per via naturale due tipi di università: da una parte un numero limitato di università di punta, in cui si fa davvero ricerca, le *Research Universities* (quali il MIT di Boston, Harvard, Berckeley, ed quali possono accedere da tutto il mondo solo gli studenti migliori, e dall'altra centinaia e centinaia di università, la cui funzione fondamentale è la buona didattica, le *Tteaching Universities*. Va anche tenuto presente che attualmente l'Italia, con poco meno dell'1 per cento della popolazione mondiale, contribuisce con la sua ricerca a non più del 3 o 4 per cento della nuova conoscenza che ogni anno viene prodotta al mondo. Per i nostri giovani e per la competitività del nostro sistema economico la cosa più importante è che tutta la nuova conoscenza prodotta nel mondo venga prontamente inserita nell'offerta formativa del sistema universitario. Occorre aggiungere che il costo dell'attività di ricerca nei settori scientifico e tecnologico è da tempo molto elevato e in continua crescita e che le risorse pubbliche per il sostegno della ricerca universitaria non possono nel nostro Paese essere ulteriormente aumentate. In conclusione, anche nel nostro Paese i tempi sono ormai maturi per avviare una ragionevole specializzazione del nostro sistema universitario, rafforzando la ricerca nelle poche università in grado di svolgerla ad alto livello, in modo da renderle sempre più competitive a livello internazionale, anche nell'attrazione di studenti da tutto il mondo, e d'altra parte favorendo al massimo lo sviluppo di una buona didattica nelle altre università, di cui non va assolutamente sottovalutata la funzione nella società della conoscenza. Come ho prima sottolineato, questa complessa transizione, di cui il Paese ha certamente bisogno, verrà avviata mediante le varie disposizioni meritocratiche nella distribuzione delle risorse pubbliche contenute nel provvedimento. nel provvedimento. Una delle innovazioni principali del provvedimento riguarda le procedure di reclutamento del personale docente delle università. Il tempo disponibile non consente di scendere nei dettagli. Vanno comunque vivamente apprezzati sia lo sforzo fatto per garantire la massima qualità e terzietà nella scelta dei nuovi ricercatori e professori, sia la decisa apertura ai giovani capaci e meritevoli, in particolare con l'introduzione nel nostro ordinamento della *tenure track*. Ne deriverà sicuramente un importante impulso al miglioramento della qualità delle attività universitarie. La struttura base del reclutamento sarà l'abilitazione scientifica nazionale. Al riguardo mi auguro innanzitutto che si riesca a mantenere elevata nel tempo la qualità scientifica degli abilitati. Non sarà una cosa facile, perché non mancheranno le pressioni per diminuire la severità dell'abilitazione. dell'abilitazione. Ogni abilitazione scientifica nazionale sarà riferita ad un determinato settore scientifico concorsuale. Sarebbe a mio avviso opportuno che il decreto ministeriale di definizione dei settori scientifico-concorsuali venisse emanato prima della conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento (non dopo 60 giorni dalla sua entrata in vigore come attualmente previsto all'articolo 13). Comprendiamo bene e condividiamo le ragioni che hanno portato all'introduzione dei settori scientifico-concorsuali. Non c'è dubbio tuttavia che l'abilitazione scientifica nazionale legata al settore scientifico-concorsuale abilita ad un ambito di discipline spesso troppo esteso. Concludo, signor Presidente, signora Ministro, prima di tutto con un ringraziamento, rivolto a tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato all'importante esame del provvedimento svolto in 7a Commissione in sede referente, durato sei mesi: ringraziamento rivolto al ministro Gelmini e ai suoi collaboratori, al relatore, senatore Valditara, ai Capigruppo della maggioranza, senatori Asciutti e Pittoni, nonché dell'opposizione, senatori Rusconi, Giambrone e Peterlini, nonché a tutti i componenti della Commissione e, naturalmente, agli Uffici della Commissione: abbiamo fatto assieme un buon lavoro. Esprimo infine, ancora una volta, un vivo apprezzamento per il testo del provvedimento al nostro esame, della cui vigorosa carica innovativa e riformatrice mi auguro le nostre università, i nostri giovani, il nostro Paese, possano presto beneficiare. Grazie Presidente, signora Ministro, colleghi, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione su un dato che è stato messo in evidenza anche recentemente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri,

dall'altra parte, la non adeguata programmazione delle immatricolazioni per quanto riguarda la facoltà di medicina e i corsi di laurea in infermieristica. So che il Ministero dell'università e della ricerca ha già cercato nell'ultimo anno di porre parzialmente rimedio aumentando i numeri. Personalmente, sono assolutamente convinta della necessità di mantenere il numero chiuso per queste facoltà, perché mi rendo conto che, oltre allo studio

soltanto in strutture ospedaliere adeguatamente predisposte; quindi i posti per avere una buona formazione devono essere adeguati.

che saremo costretti a servirci di medici che vengono dall'estero. In proposito - mi si potrebbe dire - non c'è assolutamente nulla di male, ed è così, ma allora mi domando perché ai tanti ragazzi

che tenga conto più puntualmente di tutti questi dati, eventualmente, rivaluti anche le modalità di selezione per questi corsi.

abbiamo sentito parlare molto spesso di quantità, che non necessariamente corrisponde alla qualità. Quindi, magari anche in questi pochi minuti di tempo che occuperò spero di mantenere vivo il confronto tra numeri e cose dette.

a rinsavire, di aprire le porte - pensate un po' -a persone laureate altrove, in Paesi non membri della Comunità europea, perché possano esercitare la propria professione qui in Italia, come già avviene in altri Stati membri dell'Unione europea come, ad esempio, nel Regno Unito.

questo non è stato fatto. è sicuramente un corollario, in parte necessario, in altra parte assolutamente insufficiente, di riduzione di danniaccavallatisi non negli ultimi 15 ma, mi verrebbe da dire, nei 150 anni di Italia unita, in cui non si è affrontata la questione del merito. E il merito, in questo caso, è sicuramente quello degli studenti, dei docenti e di tutti coloro i quali partecipano alla macchina amministrativa. Il primo merito, però, è quello di fare una libera scelta assumendosene tutta la responsabilità, senza entrare nell'università perché c'è bisogno di prendere tempo in attesa di trovare o un lavoro o un'altra sistemazione lavorativa - magari attraverso le maglie della politica - che possa in qualche modo aiutare a rimanere a galla. Qui dentro non c'è tutto

che secondo i radicali da sempre il problema dei problemi è l'abolizione del valore legale dei titoli di studio - affrontando, in particolare, il tema del sostegno ai nostri ricercatori attraverso la creazione ed un finanziamento congruo di un fondo premiale aggiuntivo che possa tenere conto delle professionalità, delle competenze e anche dei titoli che vengono guadagnati, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Il nostro Paese, che adesso sta delocalizzando la produzione di prodotti storici, con il passare degli anni ha delocalizzato anche la preparazione tecnico‑scientifica dei suoi cittadini, che non necessariamente provengono sempre da famiglie che siedono nei consigli di amministrazione e nei senati accademici e magari anche nelle Aule parlamentari, ma in passato ha dato la possibilità anche a chi aveva origini di tipo diverso di fare strada. Il problema è che, mentre quando delocalizziamo la produzione di automobili poi ricompriamo le vetture e ci giriamo a casa nostra, i ricercatori scientifici

i minuti necessari per affrontare nel merito la questione dell'ordine del giorno, ci tornerò magari in sede di dichiarazione di voto questo pomeriggio. Ancora una volta, però, magari rispetto ad altre situazioni dove in effetti i soldi sono necessari, si è cercato di nascondersi dietro il taglio già avvenuto, non la settimana scorsa, ma due anni fa - delle risorse necessarie alle nostre università per cancellare qualsiasi possibilità di una vera e propria riforma che non sia una ristrutturazione.

a parte la famosa scena muta, potremmo avere 322 versioni diverse di che cosa voglia dire *governance*, perché nessuno - sfido i presenti a iniziare a rispondere - sa di che cosa stiamo parlando.

prestare una particolarissima attenzione al processo che si aprirà dopo l'incontro - tutti ci auguriamo positivo, ma nessuno è in grado ad oggi di dire quanto lo sarà - che che si terrà a Torino tra il ministro Sacconi, i rappresentanti della città e i sindacati, non solo sul futuro dello stabilimento di Mirafiori, ma anche sull'attuazione del piano Fabbrica Italia. Dal processo che si apre domani a Torino dipenderà anche l'evoluzione dello stabilimento di Pomigliano e forse - data la volubilità dell'attuazione del piano FIAT - si potranno aprire o chiudere prospettive anche per lo stabilimento di Termini Imerese.

una parte del piano, a cinque anni, è focalizzata in modo specifico sull'Italia per sottolineare il fatto che le radici industriali del gruppo sono e rimarranno in Italia e che queste radici si intendono rafforzare. Continuava dicendo che Fabbrica Italia rappresenta l'impegno di FIAT per rafforzare la produzione industriale automobilistica in Italia, trasformandola in una base strategica per la produzione, gli investimenti e l'*export*. Questo era soltanto ad aprile. Le cose sembrano profilarsi, nella fabbrica globale, con difficili relazioni industriali, con opportunità ad esempio in Serbia, che non si sono schiuse negli ultimi 15 giorni (perché già il prestito BEI era stato chiesto un anno fa), in modo più problematico. Io credo che quest'Aula, con atti che naturalmente saranno congrui,